Reputo pertanto corretto portare avanti questo emendamento e mi auguro che il Governo sia favorevole.

La questione riguarda l'extragettito che non risulta inserito nell'assestamento di bilancio per l'entità dichiarata dal Governo. Vorrei sapere se è arrivata qualche indicazione da parte del Governo.

Chiedo soltanto al Governo di considerare che l'assenza del principio del contraddittorio, come d'altro canto già la Commissione affari costituzionali della Camera aveva sottolineato,

un emendamento parlamentare volto ad introdurre e modificare quel principio del contraddittorio in ottemperanza all'ordine del giorno che mi pare di capire sia la relatrice, sia il Governo hanno condiviso.

al proprio esame e chiedo al senatore Valditara, da un lato, e ai senatori Ranieri, Pellegatta e Capelli, dall'altro, se possono convergere su di una formulazione accettata da tutti, che mi pare

1-*bis* è un provvedimento assolutamente inattuabile e inaccettabile, che avrebbe reso difficile il lavoro di questa nuova agenzia di valutazione dunque sono soddisfatto del fatto che il Governo e la relatrice si siano impegnati a superare questo comma. Credo anche che la proposta di mediazione avanzata dalla relatrice sia condivisibile.

la spesa pubblica, ma indubbiamente hanno ragione i colleghi che hanno detto che, nel momento in cui si prevede un tempo pieno di qualità, occorre porre mano al finanziamento. In sostanza, non si può applicare una riforma di questo tipo

indica, come è stato ricordato, anche un piano triennale di incentivazione, finalizzato proprio al sostegno e all'incremento delle classi a tempo pieno. È un aspetto

in molte città, ad una richiesta di ampliamento della frequenza nel segmento inferiore dei primi anni della nostra scuola, a partire dagli asili nido e dalla scuola materna.

Voterò a favore del provvedimento che stiamo esaminando per le parti positive che contiene e in particolare per il tempo pieno nella scuola primaria,

il voto è positivo perché altre misure, come la valutazione dei ricercatori e le sanzioni disciplinari nei confronti degli insegnanti, che hanno suscitato tante perplessità e tante riserve, saranno riaffrontate in un quadro più organico e senza accelerazioni improprie. La necessità di un riesame è stata affermata anche dal Governo, che ha preso un impegno preciso, con nettezza, nel corso del dibattito di oggi. In particolare, è necessario collocare nel quadro di un riordino complessivo degli organi collegiali della scuola la vicenda disciplinare degli insegnanti e il proposito di disporre tutte le azioni

il dibattito di queste ore ci ha convinti di alcuni passaggi che sono che sono alla base di un documento che non ha nulla di urgente e anche di alcuni vizi di fondo che un documento come questo può avere. siamo convinti che non si tratta di un documento di urgenza: non c'è alcuna urgenza, alcun bisogno di fare le cose in fretta. Si sono fatte le cose male, come al solito si sono perse delle occasioni, ma non c'è alcuna urgenza. L'anno scolastico è iniziato

le scelte di questo Ministro, in particolare, e di questo Governo, perché sulla scuola non c'è una visione globale; si procede con decreti di questo genere o, peggio ancora, con circolari

per gli esami di maturità che non erano stati previsti. Errori clamorosi, che erano stati denunciati già in fase di riforma dell'esame di maturità; l'avevamo detto che quell'esame - che alla fine avrebbe condotto non dico non dico a niente, ma pressappoco a niente di nuovo, innovativo o utile - sarebbe stato solo un inutile costo, un aggravio di spesa. E quando i costi sono inutili, quando gli aggravi non

che pretende di essere erogatore esclusivo di un servizio e non gestore, guida di un sistema che richiede partecipazione e che in questo modo

sarà certamente accettato e non produrrà i risultati sperati e, soprattutto, non farà bene alla nostra scuola ma creerà

fare altro che respingere con tutta la forza, in attesa di poter finalmente - probabilmente fra qualche mese - assumerci la responsabilità di guidare anche questo delicatissimo settore

Signor Presidente, colleghi, vice ministro Bastico, è evidente che non avremmo approvato alcun emendamento, dati i tempi e la chiara volontà del Governo di avere questo decreto-legge approvato con rapidità. Comunque, non possiamo non esprimere apprezzamento per gli ordini del giorno accolti dal Governo, grazie ai quali si è cercato di limitare alcuni danni evidenti e colmare qualche carenza del decreto in esame; per primo, proprio il nostro ordine del giorno, che mirava ad assicurare una seria metodologia di studio del tempo pieno. Non abbiamo voluto fare inutili polemiche sui prima e sui dopo che hanno girato attorno alla problematica del tempo pieno. Eravamo e siamo del parere che il tempo pieno non può essere un modesto e dimesso tempo prolungato, un parcheggio, un tempo di custodia che garantisce qualche ora di respiro a padri e madri impegnati nel lavoro. Non ci si chiede mai se ci possono essere altri modi per soccorrere i genitori lavoratori, magari offrendo l'alternativa tra una struttura e un servizio pubblico di assistenza e la possibilità di andare in aspettativa con un assegno integrativo, tenuto conto del reddito familiare residuo. Non c'è in Italia questa possibilità di scelta presente in altri Paesi europei. Non c'è rispetto per quella famiglia che vuole educare i propri figli, che vuole tenersi in casa i propri vecchi. L'unico modello offerto e legalmente ammesso è quello del genitore lavoratore, non del genitore educatore: ci pensa lo Stato ad educare attraverso la scuola. Li vediamo tutti i giorni i risultati di questo progressivo svuotamento del ruolo educativo delle famiglie. Cari senatori della maggioranza, non saranno certo convegni, relazioni e studi sul disagio giovanile a risolvere la questione. Questi serviranno solo ad ingrassare l'immenso esercito di consulenti che gravano sulle tasche degli italiani. La realtà di un disagio giovanile così diffuso ha una sola grande radice: l'assenza della famiglia. Dobbiamo convincerci, dovete convincervi, che non tutto può dipendere dallo Stato. Moltissime famiglie in Italia assolvono il loro compito splendidamente, senza alcun aiuto dello Stato. Dovremmo essere più elastici e concepire più libertà di iniziativa da parte dei cittadini, che possono così organizzarsi in proprio i servizi necessari, dagli asili nido alle attività extracurricolari. Non dobbiamo temere questo tipo di organizzazione, anche se naturalmente sfuggirà a qualsiasi controllo da parte del potere pubblico, se non quelli per un puntuale rispetto delle leggi in materia. Per questo ho apprezzato l'iniziativa della relatrice Soliani, che accoglie il nostro ordine del giorno che impegna il Governo a potenziare nel tempo pieno attività didattiche volte ad assicurare agli alunni l'acquisizione di un metodo individuale per ottenere autonomia di apprendimento, acquisire la capacità di organizzare il proprio lavoro scolastico e utilizzare le abilità già acquisite. In pratica, la nostra preoccupazione è che mancando il classico lavoro a casa non si riesca ad imparare a studiare da soli. Quindi, non solo più tempo lontani dalle famiglia, ma anche meno seguiti, meno preparati in vista delle scuole superiori, soprattutto meno attrezzati nelle capacità di lavoro e di studio personale. Siamo anche soddisfatti perché si è sostanzialmente ripensato il comma relativo all'incompatibilità ambientale degli insegnanti. Già il termine è ripugnante. Credo che per nessun essere umano si possa dichiarare un simile stato di cose,

Non è una forma disciplinare ma cautelativa; può assumere tratti definitivi e comunque sottintende una sorta di condanna. Aver previsto almeno un serio contraddittorio è un passo avanti importante, anche in linea con il nostro emendamento. Dovremmo tornarci ancora per limitare a casi veramente unici e di grande rilevanza pubblica l'applicazione di una simile procedura. Altrimenti, sottoporremo gli insegnanti al rischio di continui giudizi, indebolendone ancora di più il ruolo ed esponendoli a metodologie giacobine nella valutazione del loro operato. Abbiamo anche approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli che porta in Commissione l'esame del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2007, con il quale si cerca di dare una risposta al problema del montante fenomeno del debito scolastico. Era il minimo che si potesse fare, vista l'evidente constatazione in base alla quale tale misura non dovesse essere adottata dal Ministro *motu* *proprio*, ma semmai inserita in un provvedimento legislativo. Siamo alle solite, onorevole Bastico. Il nostro caro ministro Fioroni crede sempre più che la scuola sia una sua questione privata e che si debba evitare il più possibile il fastidioso ricorso alla legge e al Parlamento. Bene ha fatto l'Aula, maggioranza compresa, a chiedere di discutere il provvedimento in Parlamento. Ma che sia vera discussione e non un convegno di studi nel quale il Ministro prende atto delle nostre opinioni facendole confluire in un inutile ordine del giorno, nel quale auspicheremo interventi che non saranno mai realizzati e neanche presi in considerazione. Si venga in Commissione, cara Vice ministro, aperti e disponibili ad accogliere modifiche e suggerimenti.

Quelle negative restano tutte. Il nostro Capogruppo, senatore D'Onofrio, ha opportunamente evidenziato che il decreto-legge vuole il tempo pieno ma non destina spese. Sappiamo tutti che è cosa ridicola.

Un dato è sicuro: non crescerà, né in termini qualitativi, né in termini quantitativi, senza risorse aggiuntive. Vogliamo vedere da parte del Governo in sede di finanziaria iniziative concrete. In base a quanto stanzierete per il tempo pieno valuteremo quanto crediate a questa forma di organizzazione didattica e se invece non si tratti di pura propaganda per soddisfare l'ala estrema del vostro schieramento. Vedremo quanto metterete in bilancio per finanziare iniziative per il recupero dei debiti scolastici. Da lì capiremo quanto crediate in ciò che mettete per iscritto e quanto invece sia pura propaganda. In Commissione avevo suggerito, unitamente ad altri colleghi dell'opposizione, che i grandi risparmi che si realizzeranno con il taglio di ben 47.000 docenti in tre anni vengano destinati almeno in parte per gli stipendi degli insegnanti:

Solo per dire loro grazie per quello che fanno ogni giorno sulla difficile trincea dell'educazione dei nostri bambini e dei nostri giovani. Questo poteva essere un provvedimento urgente e necessario, un primo segnale eccezionale dovuto aprire la strada ad un percorso ordinario, volto a riconoscere la specialità della loro funzione, che vogliamo affermare ancora una volta come una delle più alte missioni che lo Stato intraprende. In attesa di questi e altri segnali positivi, che per il momento non vediamo neanche enunciati, dichiaro il voto contrario dell'UDC. il provvedimento che ci accingiamo ad approvare reca disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e norme in materia di concorsi per ricercatori universitari. Esso è costituito da tre articoli e contiene provvedimenti molto eterogenei, non legati da nessi logici in sé, ma tutti accomunati dal criterio dell'urgenza, dalla volontà di mettere ordine nel tessuto della scuola e dell'università, tessuto sfinito da decenni di politiche neo-liberiste, di tagli e di marginalizzazione di ogni idea e di una pratica del sapere, dello studio e della ricerca come diritto di tutte e di tutti, come fonte di ricchezza e di benessere sociale di una nazione. Il primo problema è, dunque, il tempo e il suo rapporto con la decisione politica, le scadenze inseguite e mai compiutamente raggiunte, urgenze necessarie, che di fatto impediscono ai legislatori, al Senato e alla Camera, un dibattito ampio, articolato ed esaustivo su provvedimenti che incidono sulla qualità della scuola pubblica e dell'università. decreto, dunque, contiene luci e ombre. Le ombre si sono parzialmente dipanate nel dibattito in Commissione e in Aula, soprattutto grazie all'accoglimento di molti ordini del giorno che sostituiscono gli emendamenti che abbiamo ritirato. Alludo, in particolare, agli articoli 2 e 3, che rientrano, appunto, per noi nella linea delle ombre, della criticità e della problematicità. In particolare, tutte le disposizioni dell'articolo 2 che si riferiscono alle norme urgenti sul personale scolastico affrontano il problema di semplificare e accorciare le procedure per i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria e per il trasferimento della cosiddetta incompatibilità ambientale. Avremmo preferito discutere tutta la partita all'interno di un quadro complessivo sulla riforma degli organi collegiali e sulla valorizzazione del ruolo sociale del singolo docente e degli organismi collegiali, in cui si esercita il carattere collettivo di questa professione, sempre più complessa e difficile. L'articolo 2, a mio parere, è frutto di una fretta, giustificata ma non condivisibile, indotta dall'esposizione mediatica cui la scuola italiana è stata in questo periodo sottoposta, a partire da alcuni casi chiave, come quelli della scuola di Rignano e dal fatto che si è accettato, anche da parte delle istituzioni, di non contestare e di non contrastare la rappresentazione prevalente di una scuola pubblica ormai alle corde, attraversata e vinta dal bullismo e dalla violenza nelle aule e fuori dalle aule e da una strutturale incapacità dei docenti ad esercitare la loro funzione di educatori, di maestri, capaci di trasmettere conoscenza, sollecitare intelligenza, passione per il sapere capacità di attraversare il mondo con uno sguardo critico. Non era necessario partire da qui. Questo partire da qui è sentito come un giudizio di valore negativo su tutto il corpo docente. Per questo è importante che nell'articolo 2 si richiami in continuazione il rispetto per la libertà dell'insegnamento e per l'autonomia dei docenti, a testimonianza del fatto che la materia su cui ci si muove è un crinale difficile e che ci confrontiamo su norme oggettivamente transitorie perché parziali ed emergenziali. Anche l'articolo 3, in particolare al comma 1-*bis,* ci vedeva in netto dissenso. Nonostante nella passata finanziaria

che ne consente la nascita, sulla sua missione e sul suo funzionamento), si era partorita una norma con un doppio difetto: da un lato, vi era una discriminazione che avrebbe fatto dei ricercatori neo-assunti i primi e i soli soggetti valutati individualmente dall'Agenzia, senza che questa operazione si dilatasse a tutti i livelli della ricerca e della docenza; dall'altro - e questo è l'elemento più grave - si consolidava un'idea della funzione dell'Agenzia come valutatrice dei singoli e non del sistema. Ma il decreto, dicevamo, contiene anche una luce, strutturale e importante, ed una positività prevalente, che ci inducono ad esprimere un voto ampiamente positivo: si tratta dell'articolo 1, l'unico che ha valore ordinamentale e duraturo. Questo articolo unico ripristina il tempo pieno, il tempo prolungato, nella sua forma originale premorattiana: si raccoglie, insomma, l'istanza di un vasto movimento che ha animato le scuole di passione pedagogica e partecipativa, che ha unito genitori e docenti in una nuova modalità di collaborazione e di partecipazione democratica, che ha ricollocato nella contemporaneità il tempo pieno, quel modello pedagogico e strutturale della scuola italiana di base che per decenni ne ha garantito la qualità, rispettando la centralità dei bambini e delle bambine, relazionandosi alle loro vite concrete e intrecciando con le famiglie relazioni ben più strette di quelle formalmente sancite dagli organi collegiali. Tempo pieno, quindi 40 ore, ore di compresenza, due docenti: questo è il tempo pieno che viene ripristinato, ma l'articolo 1 supera gli stessi limiti del testo unico che aveva sancito questa forma. Rispetto ai tetti degli organici degli anni 1988 e 1989, questi tetti vengono cancellati e s'impegna il Governo, di concerto con le Regioni, ad elaborare un piano di espansione e di promozione del tempo pieno su tutto il territorio nazionale. Le 40 ore della Moratti non erano nel tempo pieno, non c'erano due insegnanti, c'era lo spezzatino delle ore, c'era una scuola che non aveva questo tempo lungo disteso, ma obbligava i bambini a passare da un insegnante all'altro e a non avere i loro insegnanti di riferimento: era un'altra cosa. Non bastano le 40 ore: ci vogliono le 40 ore, due insegnanti e le ore di compresenza, nelle quali si può fare quello che alcuni che alcuni ordini del giorno chiedono (cioè quel lavoro individuale di abitudine alla riflessione che molti falsamente pensano non si possa fare frequentando il tempo pieno). Altri lati positivi sono il ripristino dell'ammissione agli esami di terza media da parte del consiglio di classe, a indicare il rigore e la serietà che si vogliono attribuire a questa prova, come pure la disposizione positiva che carica il Ministro dell'economia al pagamento delle supplenze per maternità

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci troviamo dunque ad esprimere un voto su questa finta riforma Fioroni.

«disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico», abbia già *in* *nuce* una sua dichiarazione di fallimento. Ritengo che la disciplina di un ordinato avvio debba essere varata, approvata ben prima dell'avvio stesso. E, non a caso, questo provvedimento giaceva alla Camera dal febbraio di quest'anno. Devo anche aggiungere che, nonostante la buona volontà dimostrata dal Sottosegretario nel cercare di difendere questo provvedimento, non ha risposto alla mia prima osservazione, al fatto che questo provvedimento non ha consentito comunque di evitare quelle inefficienze gravi che hanno caratterizzato l'avvio dell'anno scolastico nel nostro Paese. Ho denunciato e voglio qui ribadire il fatto che, in queste settimane, i nostri ragazzi, i nostri giovani si sono trovati di fronte ad una miriade di insegnanti supplenti che cambiavano di giorno in giorno di fronte a cattedre scoperte come mai era avvenuto negli ultimi sei anni. È dunque una dichiarazione certamente di fallimento. Voglio, però, anche aggiungere che pure le parole della relatrice Soliani, che apprezzo per l'onestà intellettuale che ha dimostrato, testimoniano come non vi sia, da parte della relatrice di questo provvedimento, una sostanziale condivisione del metodo, dell'impostazione della politica scolastica di questo Ministro. E veniamo ad alcuni punti su cui la posizione del Governo non è stata affatto convincente e che dunque inducono Alleanza Nazionale a votare convintamente contro questo provvedimento. Il tempo pieno. il tempo pieno è in realtà un clamoroso inganno: l'ho già detto in discussione generale. ribadire all'onorevole Sottosegretario che le famiglie vogliono le 40 ore e noi le avevamo garantite. Anzi, voglio qui aggiungere che nella passata legislatura le classi a 40 ore erano persino aumentate. Non credo che le famiglie italiane vogliano le compresenze. Le compresenze le vuole un certo sindacato, la CGIL, per esempio, per aumentare a dismisura l'organico degli insegnanti, dunque per sprecare risorse anziché concentrarle nella valorizzazione professionale degli insegnanti. Così come anche credo che il tempo pieno non serva per garantire un migliore inserimento degli alunni stranieri. Alleanza Nazionale ha fatto una proposta molto precisa nel suo disegno di legge di riforma organica della scuola: *test* di ingresso di lingua e, nell'ipotesi di mancata conoscenza della lingua italiana, corsi obbligatori organizzati dai Comuni con il contributo dello Stato per consentire a questi giovani di potersi inserire pienamente nelle nostre scuole. Perché, cari colleghi, quando un ragazzo di 12-13-14 anni od anche più viene inserito in una scuola senza conoscere una parola d'italiano,

c'è il pagamento delle supplenze sottolineato in alcuni interventi: qui c'è stato veramente un clamoroso *flop* della politica scolastica di questo Governo che, a partire da febbraio,

per cui i ragazzi di fronte ad un insegnante che si ammalava venivano spostati da una classe all'altra o addirittura invitati a rimanere a casa perché non vi erano i soldi per le supplenze. E questo per via di un provvedimento contenuto nella scorsa finanziaria voluto da Padoa-Schioppa/Fioroni, un provvedimento in base al quale voi avete scaricato sui bilanci delle scuole gli oneri della della gestione delle supplenze. Ora, in ritardo rimediate ad un vostro clamoroso errore. L'esame di Stato. Ho qui i dati. La percentuale di non ammessi a seguito dello scrutinio è pari al 4,4 per cento. La stragrande maggioranza dei maggioranza dei "bocciati" dalla nuova maturità è dovuta alla reintroduzione dello scrutinio di ammissione che venne abolito da Berlinguer e venne già reintrodotto dalla Moratti, sospeso e cancellato da Fioroni e poi reintrodotto da Fioroni. E allora, nulla di nuovo, se non un onere aggiuntivo particolarmente rilevante a carico dei bilanci delle scuole italiane La valutazione delle scuole. Abbiamo perso un anno e mezzo: era già previsto dal passato Governo; è stato reintrodotto alla Camera grazie ad un emendamento dell'opposizione.

Si è dimenticato, cioè, di inserire nel nostro sistema scolastico principi che riportino al centro della scuola la figura del docente, che ridiano autorevolezza all'insegnante e che, soprattutto, ripristinino il principio di autorità nelle nostre scuole.

facendo mancare alle università e alla ricerca italiana per un anno i finanziamenti (rimanendo dunque a secco la ricerca italiana); è arrivato tardi sull'Anvur, lo abbiamo denunciato oggi è arrivato tardi, anzi non è arrivato ancora per nulla, sui concorsi per associato e per ordinario (altro che dare spazio ai giovani!); arriva tardi sui ricercatori ripristinando le vecchie regole che nella scorsa finanziaria aveva dichiarato di voler abrogare,

Sull'ANVUR e sulla valutazione dei ricercatori l'opposizione ha vinto: avevamo dichiarato in Commissione che se il nuovo organismo di valutazione avesse dovuto valutare gli articoli e i libri di migliaia di ricercatori francamente non sarebbero bastati dieci anni.

chiedendo che in un prossimo urgente provvedimento il Governo cancelli - perché sostanzialmente la revisione è una soppressione - questa norma. È una vittoria - ripeto - dell'opposizione.

mesi, non più soltanto la riedizione in forma riveduta e corretta della riforma Moratti, ma risposte chiare su alcuni temi scottanti. Intanto, la reintroduzione del merito: chiedo, per esempio, che gli stipendi dei docenti possano essere in qualche modo commisurati anche ad una valutazione meritocratica. Infine, come già accennavo, la reintroduzione di un principio di autorità: per esempio,

Responsabilizziamo le famiglie! Insomma, si tratta di superare il modello di scuola del '68 per ripristinare una scuola seria, formativa, che dia un avvenire certo ai nostri giovani.

Signor Presidente, colleghi senatori, è sotto gli occhi di tutti che l'avvio dell'anno scolastico 2007-2008 presenta alcuni problemi procedurali dovuti in parte alla rapida successione di disposizioni che in questa materia sono state apportate negli ultimi anni. È altrettanto evidente che la legge di conversione che ci apprestiamo a votare provvede a risolvere alcuni di questi problemi, primo fra tutti tutti la reintroduzione nella scuola primaria delle classi a tempo pieno, una disposizione adottata, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, per venire incontro alla crescente domanda delle famiglie italiane di progetti formativi a tempo pieno o prolungato che abbiano l'obiettivo di ampliare il bagaglio culturale degli alunni. Altro pregio che possiamo senza alcun dubbio attribuire a questa legge è di iniziare a razionalizzare metodi e procedure che avevano generato abusi e disfunzioni, come nel caso delle procedure per gli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado, per le quali sono state introdotte norme più rigorose per l'individuazione della sede di esame per i candidati esterni. Viene inoltre innalzato di 45 milioni di euro - portandolo a 183 milioni il limite massimo di spesa per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria, aumento di spesa che servirà ad adeguare dignitosamente i compensi dei membri delle commissioni d'esame. Altra disposizione molto importante è quella che dispone, per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, che vengano riconosciuti come titoli abilitanti all'insegnamento anche i diplomi conseguiti presso gli appositi istituti, per i docenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge n. Sono solo alcune delle norme più qualificanti di questo disegno di legge, che sicuramente non risolverà per intero e una volta per tutte gli atavici problemi della nostra scuola, ma che certamente rappresenta un grosso passo in avanti per mettere in linea e rendere competitivo il nostro sistema scuola con quello degli altri Paesi europei. La cultura rappresenta per i nostri giovani un imprescindibile pilastro in vista delle sfide del futuro ed al tempo stesso un baluardo, anzi il fondamento stesso della democrazia: su questo non è possibile pensarla diversamente.

nel dichiarare il voto dei senatori che aderiscono alla costituente socialista, vorrei ricordare al Governo e all'Aula che i parlamentari socialisti alla Camera

un insegnante ad assolvere alla sua professione. L'aver sottoposto gli insegnanti alla potenziale gogna del giudizio dei familiari un presupposto che non possiamo accettare, fa parte di un altro modo di concepire la scuola, il rapporto con il mondo della scuola e l'autonomia dell'insegnamento. Per tale motivo vogliamo sottolineare questa nostra esplicita riserva. Avremmo voluto astenerci dal voto. Non lo facciamo

l'altro ieri ma all'inizio della legislatura. È bravissimo a fare esternazioni, è bravissimo a inventare parole, è bravissimo a raccontare balle

Dico questo, Presidente e signori colleghi, e vi ringrazio di ascoltarmi e per la vostra gentilezza, perché sulla scuola si fa un gran parlare, ma nella scuola crescerà o non crescerà il futuro della nostra società. Ebbene, se si continua a governare come oggi governano il ministro Fioroni e questa maggioranza, uccideremo

si mette in condizione, questo Governo, questo Ministero, di adottare forme più repressive nei confronti degli insegnanti. In virtù di che cosa? In virtù dell'effetto Rignano: c'è la contingenza, perché alcune famiglie hanno messo all'indice alcuni insegnanti. Si dà in mano ad un solo personaggio, che è il direttore scolastico, il potere, senza nemmeno avere il contraddittorio, di allontanare o meno un insegnante.

ed il fatto stesso che il Governo abbia accettato numerosi ordini del giorno che lo impegnano a rivedere questo decreto-legge la dice lunga sul fatto che quel che sto dicendo è pura verità. Parliamo Parliamo dell'iniziodell'anno scolastico regolare. Dopo cinque anni di Governo del centro-destra, il primo anno in cui non è regolare l'inizio dell'anno scolastico è proprio sotto il Governo del centro-sinistra. Stanno ancora mancando insegnanti: nella stessa Roma, capitale d'Italia, ancora non ci sono gli insegnanti. Questa è la realtà, altro che buon inizio dell'anno scolastico! tempo pieno, ci stiamo prendendo in giro ancora una volta, perché basta rileggere il dispositivo, che recita: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Cara senatrice Capelli, capisco che vorresti gioire di questo, ma per gioire devi trovare le risorse per la doppia presenza in classe degli insegnanti, perché dove trovi gli insegnanti, se non hai i denari per portare avanti il tempo pieno? In realtà, quindi, è di nuovo un proclama messo in legge, che nello stesso tempo la legge annulla, perché non deve gravare sulla finanza pubblica e i fondi non ci sono. Tant'è, che il Governo si è impegnato e ha accettato l'impegno a trovare i soldi in finanziaria. Aspettiamo, vedremo se troveranno, se troverete i soldi nella finanziaria.

i ricercatori, ma solo i ricercatori, perché i professori associati e ordinarinon si toccano. Valutarli poi come? Con una struttura, caro Presidente, che ancora non esiste: l'ANVUR.

Bene, questo Governo è capace anche di trasporre in legge qualcosa che non esiste: l'ANVUR. Veramente c'è tanto da ridere! È di questi giorni il proclama, di nuovo, del ministro Fioroni: «più serietà».

I debiti vanno recuperati giorno per giorno, periodo per periodo, non dopo uno, due o tre anni, perché non si recuperano più. Lo sapete voi e lo sappiamo noi, dobbiamo avere il coraggio di dirlo!

il problema educativo si recupera parlando con le famiglie, parlando con gli insegnanti, tornando a dare dignità alla funzione docente. *(Applausi dal Gruppo FI).* Se non si torna a dare la vera dignità alla funzione docente, il loro impegno non c'è, l'educazione non esiste e non si cresce. In conclusione, signor Presidente, con questo Governo, ma soprattutto con il ministro Fioroni, abbiamo scoperto una cosa: non riusciamo, né noi dell'opposizione ma nemmeno voi della maggioranza, a capire cosa abbia in testa quell'uomo, come vuole la scuola, qual è il quadro normativo, dove la vuole ricondurre, quali sono le sue direttive! Non ci sono, non ha idee, ha solo *slogan*, solo *slogan*, solo *slogan*! Ebbene, con questi *slogan*, signor Presidente, Fioroni andrà a casa, spero quanto prima, assieme a tutto il Governo di centro‑sinistra. trovo qualche contraddizione tra il dibattito sereno, di merito, che svolgiamo in Commissione e che trova sbocco in ordini del giorno ampiamente unitari, in cui maggioranza e opposizione ragionano concretamente sul provvedimento e indicano anche i correttivi necessari, e - permettetemi, colleghi - il tono un po' propagandistico che assume la discussione in Aula. Credo che la scuola italiana abbia bisogno di serenità

stabilire se i provvedimenti sono più o meno distanti dalla riforma Moratti o da qualcos'altro: i provvedimenti vanno valutati nella loro concretezza e per la loro capacità di rispondere ai problemi della scuola italiana.

venga ripristinato, così come l'avevamo pensato, così come l'aveva voluto la parte migliore della scuola italiana, non - mi permetta, senatore Marconi per indebolire il ruolo educativo delle famiglie, ma per impedire in qualche modo che il successo e l'insuccesso scolastico in questo Paese dipendesse dalla condizione socio-culturale della famiglia d'origine,

che servisse ad attenuare le differenze che provenivano dalle condizioni socio-culturali delle famiglie d'origine. Quanto alla questione delle famiglie, vorrei che ne discutessimo una volta seriamente. Lo schema che mette la famiglia contro la scuola, «più scuola, allora meno famiglia», «più funzione educativa dello Stato, meno delle famiglie», permettetemi, non funziona proprio. Noi viviamo una drammatica crisi educativa delle famiglie,

di spontaneismo, senza valori, e l'atteggiamento del genitore verso la scuola è quello di fare il sindacalista del proprio figlio. Questo è un problema di tutti e e studiare e lavorare su nuove forme di partecipazione e di intreccio tra scuola e famiglia rappresenta il modo migliore per dare la risposta giusta. Ma dobbiamo lavorarci insieme, senza che nessuno assuma

con questo provvedimento, ci sarà una maggiore responsabilizzazione della scuola rispetto alle supplenze. Sono contento perché c'è una norma che gli oneri derivanti dalle supplenze di maternità a carico di un fondo ministeriale per i contratti a tempo determinato. La trovo una previsione importante. Chi vive nella scuola lo sa: i dirigenti scolastici possono organizzare meglio il lavoro, per ricorrere meno alle supplenze, non possono organizzare la politica demografica del Paese. E quindi, il fatto che il Governo centrale costituisca un fondo per la supplenza di maternità, dotandolo di 66 milioni

vuol dire costruire un progetto organico che in qualche modo costringa le università a rendere conto di chi assumono

È successo in questi anni, con il ministro Moratti, e probabilmente anche con i Governi precedenti. Allora, con questo provvedimento si afferma una cosa chiara: le scuole devono dire quali strumenti mettono a disposizione dei ragazzi per recuperare i debiti e valutare se li hanno recuperati a partire dal lavoro che essi hanno fatto. La scuola che valuta se hanno recuperato oppure no i debiti è quella che deve dimostrare di aver messo in atto gli strumenti perché i debiti siano recuperati.

e, quindi, si stabilisce anche sulla base della variazione delle richieste delle famiglie. Lo verificheremo, ma questo è quello che c'è scritto. Non c'è scritto che il tempo pieno si fa comunque, ad organico invariato: si stabilirà anno per anno, sulla base delle richieste, ciò che è necessario attivare. In secondo luogo, non c'è un organico distinto del tempo pieno: l'organico del tempo pieno è quello che deriva dall'organico complessivo. detto tutto questo, con molta serenità, noi non votiamo un provvedimento che risolve i problemi della scuola italiana, ma un provvedimento che rende la scuola italiana un po' più serena, che le mette più strumenti a disposizione, che le toglie un po' d'ansia. Questa è stata l'attività complessiva del Governo in questo anno e mezzo. Vi farà piacere oppure no, ma la scuola italiana sembra un po' più serena di quella del tempo della Moratti; e non è più serena perché gli insegnanti sono tutti comunisti e quando c'era la Moratti facevano casino - scusate il termine - e adesso che c'è Fioroni stanno tutti bravi: sono più sereni perché trovano un Governo

parte da una constatazione, cioè che questo provvedimento è un autentico attacco illiberale e autoritario alla libertà d'insegnamento, penso non si possa esprimere in due minuti. rimanere agli atti dell'Aula che in questo Senato si vota un nuovo articolo 468 che prevede il trasferimento per incompatibilità ambientale. Probabilmente, molti colleghi non hanno capito bene di cosa si tratta. È detto in questo articolo che «il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico», ricorrano ragioni d'urgenza. Ma non basta: «Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti Quindi, viene sollevata l'incompatibilità e il provvedimento di sospensione del docente, in questo caso, avviene «senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1» di questo

scolastico, una norma illiberale, autoritaria e dispotica come questa, senza rendersi conto, né la maggioranza né l'opposizione, di quello che si va a votare, ritengo, per dignità mia personale, di astenermi dal voto e uscire dall'Aula.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 26 settembre scorso ha avuto luogo la votazione degli articoli del rendiconto e che nella seduta pomeridiana del 2 ottobre ha avuto inizio la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di assestamento.

esso, alla pari di altre impostazioni dell'assestamento come la diminuzione dei trasferimenti all'Unione Europea, sembra finalizzato non a rendere

in relazione all'andamento dell'economia nel resto dell'anno, ma semplicemente a coprire un decreto-legge che trae da presunte entrate motivi per allargare i cordoni della borsa e fare una specie di spesa che, congiuntamente alla finanziaria, non ha altre caratteristiche di una improvvida spesa elettorale, quando invece si sarebbe dovuto risparmiare e conseguire risultati nel contenimento della spesa pubblica, come ci insegnano all'interno la Banca d'Italia e la Corte dei conti, all'esterno il Fondo monetario e

Dichiaro aperta la votazione.

precisare che gli elementi di risposta che fornirò ora all'Aula sono stati dal Governo, nella mia persona, rappresentante*pro tempore*, forniti in Commissione bilancio, allorché un simile quesito era stato sollevato dal senatore Baldassarri. Quindi, non è vero che il Governo non ha fornito una risposta: la risposta era stata a suo tempo fornita nella 5a Commissione permanente, allorché vennero approfonditi questi temi. Il senatore Baldassarri sostiene che vi sia incongruenza tra i dati rivenienti dall'analisi degli incassi tributari del bilancio dello Stato, il cui assestamento quest'Aula si si accinge ora a votare, e i dati relativi al conto economico delle amministrazioni pubbliche, che si ritrovano, tra l'altro, in documenti quali la Relazione previsionale e programmatica e il Documento di programmazione economico-finanziaria. Ebbene, il confronto che fa il senatore Baldassarri affermando che nel bilancio dello Stato appaiono incrementi per 12 miliardi, mentre nei documenti relativi alla pubblica amministrazione

diversi tra loro. Il bilancio dello Stato, come ovvio, riporta l'andamento degli incassi tributari dello Stato. Il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, oltre agli incassi tributari dello Stato, riporta altre voci di entrata, quali, ad esempio, all'interno degli stessi tributi erariali, la parte che afferisce al bilancio delle Regioni a Statuto speciale; in secondo luogo, i tributi propri di Regioni, Province e Comuni, che ovviamente non possono essere inclusi nel bilancio dello Stato, così come l'andamento dei contributi sociali, incluso nel conto economico della pubblica amministrazione ma che ovviamente non può essere incluso nel bilancio dello Stato; e, da ultimo, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione vi sono i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. È quindi del tutto evidente che le due grandezze siano completamente separate, nel senso che i dati riportati nel bilancio dello Stato sono una parte, ancorché modesta, del totale delle entrate che si evince dal conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Pertanto, un confronto tra la variazione operata in corso d'anno nel bilancio dello Stato e la variazione operata in corso d'anno in documenti ufficiali relativi al conto economico consolidato non può assolutamente essere fatto. Si può stabilire un raccordo tra le due, ma non si può affermare che la prima variazione debba essere uguale alla seconda, per i motivi che spero siano ora del tutto ovvi e che erano stati

tra accertamento e assestamento: l'accertamento è un atto amministrativo obbligatorio attraverso il quale si accertano maggiori entrate via via che le stesse afferiscono al bilancio dello Stato; l'assestamento si riferisce al bilancio dello Stato ed è un atto che può essere discrezionale. Pertanto, ciò che conta ai fini della copertura di un provvedimento non è l'assestamento ma è l'accertamento, che è già avvenuto da tempo.

ma la mia domanda non era riferita, ovviamente, alla differenza tra il bilancio dello Stato e il bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, ma semplicemente la domanda resta e non ha avuto risposta - a ciò che il sottosegretario Sartor ha appena accennato. La mia domanda era: qual è il il quadro di coordinamento che porta il Governo a sostenere che ci sono 19 miliardi in più nel bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni e soltanto 12 miliardi di euro in più nel bilancio dello Stato? Qual è tale raccordo? Questa era la richiesta e non volevamo che ci spiegasse la differenza tra bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti territoriali e non territoriali che nel bilancio afferiscono al bilancio delle pubbliche amministrazioni, materia nota a qualunque studente di primo anno di scienza delle finanze; almeno ai miei tempi

ha dichiarato che il maggior gettito di quest'anno è pari a 25 miliardi di euro nel bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni?

a fine settembre. Allora, l'altra questione è: se il Governo ha dichiarato 25 miliardi di euro di maggior gettito nel bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni,

supposto. Il fatto che sia auspicato è un di più rispetto alla previsione regolamentare. Il problema di oggi, signor Presidente, non è verificare il numero legale per essere confortati rispetto alla necessità di una presenza usuale, ma è quello di accertare una presenza eccezionale, perché stiamo votando parti fondamentali

non soltanto per ragioni di tipo tecnico (per quanto possa esserci qualcosa di tecnico nella politica economica) o per motivi politici (per quanto non vi può essere proprio nulla di politico che non sia anche tecnico in politica economica). Non lo siamo per il particolare motivo

cercato di convincerci che l'uno non è l'altro. Tuttavia, è pur certo - come ricordava il collega Baldassarri - che l'uno dinamicamente dovrebbe cercare di correggere l'altro e quando l'uno e l'altro presentano così profonde differenze, come quella che si realizza nelle letture contabili, ne deriva una notevole perplessità.

di incrementare le risorse disponibili per la trattativa sul *welfare*). Tralasciamo il fatto della corrispondenza della cifra e della contemporaneità delle decisioni adottate per dire che, d'altro verso, i nostri emendamenti sono presentati nel tentativo di correggere le tabelle correttive presentate dal Governo in un modo che riteniamo essere migliorativo rispetto a quelle stesse correzioni.

del FAS per poi utilizzarle nel decreto-legge n. 159 (collegato meccanicamente, anche se non secondo le leggi di contabilità, alla manovra finanziaria) e, contemporaneamente, ancora, vendersi, nelle tabelle della finanziaria futura, che i fondi per il Mezzogiorno aumentano, sino ad arrivare a 100 miliardi a 100 miliardi nei prossimi quattro anni, mentre, allo stesso tempo, gli ultimi tre o quattro mesi di quest'anno vedono una decurtazione notevolissima di un miliardo

una cassa che piange e, quindi, non si fanno i trasferimenti alle Regioni, agli imprenditori, a coloro che hanno compiuto gli investimenti o hanno assunto per i decreti che li autorizzavano agli impegni di spesa; dall'altro, si tagliano le disponibilità, creando una difficoltà globale nel sistema Paese. Infatti, da un lato, si promette di dare e, dall'altro, invece, non vi è alcuna elargizione immediata, anzi, c'è un taglio che cerchiamo di correggere: tutto questo lascia intravedere una

pubblica amministrazione con quelli del bilancio dello Stato e che, però, vi è una tavola di raccordo. Allora, vorrei capire se il Governo intende fornire all'Aula del Senato questa tavola di raccordo oppure no. no. Posso testimoniare - in forza dei cinque anni trascorsi al Ministero dell'economia in qualità di Vice ministro - che la Ragioneria dello Stato fornisce regolarmente al Gabinetto del Ministro dell'economia la tavola di raccordo tra la pubblica amministrazione ed il bilancio dello Stato. Quindi, questa tavola esiste perché l'Aula del Senato non può essere a conoscenza di questi numeri; esiste anche la tavola di raccordo tra cassa e competenza, proprio perché sono definizioni radicalmente diverse. Dunque, signor Presidente, vorrei che il Governo rispondesse in Aula se intende spiegare (il più rapidamente possibile

del consolidato delle pubbliche amministrazioni ai 12 miliardi del bilancio dello Stato. È una tabella che - ve lo garantisco - esiste e non può rimanere nascosta nei cassetti segreti della Ragioneria dello dello Stato né di quelli del Gabinetto del Ministro. È l'Aula del Senato che deve essere a conoscenza di questi dati. *(Applausi

mi scusi ma il mio posto era stato momentaneamente occupato dal collega Piccone. Noi cerchiamo di intervenire sulla Tabella 2

al Paese come una migliore attenzione rispetto alle libertà civili e a quelle dell'immigrazione. C'è la necessità di intervenire nel campo forestale e rileviamo che il Governo ad un utilizzo insano delle risorse disponibili. Nell'assestamento viene corretta la cifra del saldo netto da finanziare con riferimento ai 7 miliardi

tra l'utilizzazione delle risorse prevista prima del periodo feriale, le necessità che si sono rilevate durante il periodo feriale e quanto invece non si è prodotto né nell'assestamento, né nei provvedimenti all'esame dell'Assemblea.

Presidente, mi perdoni, ma dato il silenzio del Governo dobbiamo prendere atto che questa Assemblea procederà a votare il bilancio di assestamento senza conoscere i numeri. O no? Vorrei poter essere smentito. Il Governo intende fornire questa Tabella di raccordo? Vorrei sentire un bel "no", forte e chiaro, da parte del Governo. PRESIDENTE. Può darsi che questa volta chi tace dissenta e non acconsenta.

che non si possono ricondurre a condizioni di sicurezza perché non esistono le risorse necessarie. Allora, come non pensare di voler dare anche un piccolo significato di volontà del

dei 50 milioni in più all'Istituto Gaslini di Genova o ai 150 milioni alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la bretella di collegamento autostradale di Trieste. Si approvano, cioè, degli interventi puntuali ma che hanno la caratteristica di una manovra espansiva assolutamente non condivisibile, e, quando invece si parla di implementare le risorse per un comparto

per l'organizzazione giudiziaria e per le esigenze di mantenimento dei compiti di difesa, auspichiamo che l'attenzione dei colleghi e della maggioranza sia massima.

di legge di assestamento è un provvedimento formale, ma non c'è formalità che si ricolleghi ad un bilancio e ad una finanziaria precedenti che hanno un significato specificatamente politico che possa essere tale; ha una formalità nel senso che si riferisce a numeri, a correzioni.

Presidente, mi consenta di intervenire per una richiesta relativa ai mezzi operativi e strumentali del Corpo forestale dello Stato, anche

L'emendamento 1.2 è stato dichiarato inammissibile perché il bilancio di assestamento è considerato una operazione formale e non può introdurre decisioni di sostanza.

di due cose fondamentali: la prima, è che l'Assemblea del Senato vota un bilancio dello Stato senza conoscere perché vengono apportati certi numeri; la seconda, è che si considera un assestamento formale, al di là della diversità dei numeri, un assestamento che cambia le entrate dello Stato per 12 miliardi di euro, cioè 24.000 miliardi di vecchie lire. Questo è considerato un mero aggiustamento formale, di cui ero primo firmatario, viene giudicato inammissibile per aspetti puramente giuridici. Signor Presidente, vorrei semplicemente segnalare ai colleghi

dei cittadini meno fortunati del nostro Paese, che l'emendamento 1.2 consiste nell'abrogare il cosiddetto

dispersi in 30 voci diverse e messi a discrezione dei Ministri. Ebbene, l'emendamento 1.2 proponeva di assegnare quelle risorse

che invece di dare 81 centesimi al giorno ai pensionati minimi si propone di dare loro 120 euro al mese, togliendo tale somma dalle grinfie e dai cassetti segreti dei Ministri di questa Repubblica e mettendola direttamente nelle tasche delle persone che ne hanno bisogno: i vostri pensionati minimi.

con la vergogna dei vostri 81 centesimi, per mettere poi gli altri cinque miliardi di euro nel bilancio dei vari Ministeri dispersi in mille rivoli, e l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa a parità di risorse, senza un euro in più di *deficit*, al contrario di quanto ha fatto il Governo che quest'anno

Questo è il giudizio di inammissibilità sull'emendamento 1.2, quando nella sostanza veramente inammissibili - o meglio, inaccettabili - sono un Governo che nasconde i numeri e una maggioranza che fa finta di non saperlo, pur di far sopravvivere qualche giorno o qualche settimana

che il raccordo cui si riferisce il senatore Baldassarri riguarda il conto economico consolidato dell'amministrazione pubblica, non il bilancio dello Stato. Tutti gli elementi informativi necessari per poter votare con piena cognizione di causa sono contenuti, come è ovvio, nel documento di bilancio che è all'attenzione dell'Aula e nei relativi emendamenti riferiti agli assestamenti. Quindi, non vi è alcuna omissione di dati o di informazioni, quale che sia. Il voto - è ovvio che sia così - si esprime su un documento trasparente e rispettoso. Per quanto riguarda la presunta tabella di raccordo relativa al conto economico della pubblica amministrazione, direi che innanzitutto è sufficiente leggere con attenzione le tabelle incluse nel Documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento - ribadisco - al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, laddove si troveranno analiticamente indicate non solo la voce relativa agli incassi tributari, ma anche le voci relative all'andamento degli introiti per contributi sociali obbligatori e per altre entrate quali i proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Quindi, non vi è bisogno di alcuna tabella di raccordo, ma è più che sufficiente un'attenta lettura delle tabelle che già sono state offerte a quest'Aula, al Parlamento in generale e alla pubblica opinione. Pertanto, non vi è bisogno di nulla se non di un'attenta lettura. La improponibilità del raffronto cui facevo riferimento non è tra bilancio dello Stato e conto economico. Come ho ribadito nel mio intervento, il bilancio dello Stato rappresenta il di cui di una parte molto più grande, che è il conto economico, ma è assolutamente improprio confrontare le variazioni delle entrate riportate nel bilancio dello Stato con le variazioni riportate nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

attenzione. Per quanto riguarda il conto economico, lo sono da ancora più tempo, nel momento in cui sono stati presentati il Documento di programmazione economico-finanziaria e la relativa Nota di aggiornamento. Ciò che è richiesto è semplicemente un'attenta lettura delle tabelle che sono ivi incluse.

Il senatore Baldassarri ha chiesto alcuni dati, per spiegare alcune incongruenze che a lui sembra di rilevare fra il conto economico della pubblica amministrazione e il bilancio che è sottoposto alla nostra approvazione. Il Governo, che non ascolta ciò che si dice nell'Aula, confermando con ciò l'atteggiamento di profondo disprezzo che nutre nei confronti FI)*, ci ha dato una lezione di scienza delle finanze, spiegandoci la differenza tra conto economico e bilancio dello Stato. Voglio rassicurare il signor Sottosegretario che tale differenza è nota anche ad un povero filosofo come me immagino ancor di più ad un cattedratico di economia come il collega Baldassarri), dalle memorie delle lezioni del professor Cosciani, quando frequentavo la Facoltà di giurisprudenza qui a Roma.

analiticamente, di cosa si tratta, come mai emerge e cosa la giustifica. In seconda battuta, il signor Sottosegretario ci dice che questi dati sono deducibili da altro documento a disposizione.

quest'Aula quantitativamente, non per elencazione di voci, ma per elencazione di quantità corrispondenti, a cosa corrispondono questi atti. Il Governo vuole dircelo? Prima di poter votare con piena coscienza, riteniamo di avere bisogno di questi dati. Il Governo intende sindacare una domanda di informazioni fatta dal Senato? Ritiene di non avere il dovere di rispondere? Ci dice che questi dati non sono attinenti al bilancio.

un secondo mistero: il preconsuntivo del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2007, dopo che il Governo ha dichiarato che c'era un extragettito di 25 miliardi,

lo scorso anno): quest'anno (nel 2007) le pubbliche amministrazioni incassano 728 miliardi di euro,

che da 728, il tendenziale del 2008 automaticamente verrà sottostimato dal Governo, che nasconderà alla sua stessa maggioranza il dato vero sulle risorse disponibili, in attesa di scoprire, da marzo 2008 in poi, nuovi tesoretti. Quest'ordine del giorno impegna il Governo ad indicare il numero vero per il 2007;

e sanità», svolta dal Ministero della salute. Alcuni giorni or sono, in una trasmissione televisiva, la Ministra, interpellata dal collega Mantovano, non ha saputo spiegazioni sui costi di questa campagna, attualmente in vigore. Potrei fare una battuta, chiedendo se l'ha copiata del vecchio De Sica («Pane, amore e fantasia»), ma non è questo il problema. Il problema di fondo è che la campagna è attuale. Le chiediamo

una risposta urgente del Ministro dei trasporti sull'avviata procedura di soppressione dell'autorità portuale di Trapani. Inopinatamente il Ministro, non tenendo conto di questo e di altri atti di sindacato ispettivo presentati anche alla Camera, ha mandato avanti quella procedura, sottoponendo alla firma del Capo dello Stato il provvedimento di soppressione, palesemente illegittimo e privo del concerto del Ministro delle infrastrutture e dell'intesa del Presidente della Regione siciliana. Quindi preannuncio che, ove

ma ha ritenuto di bypassare accelerando procedure che, invece, proprio in considerazione dell'esistenza di atti di sindacato ispettivo a firma di tutte le forze parlamentari, di maggioranza e di opposizione, avrebbe dovuto, quanto meno, sospendere.